finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

Signor Presidente, colleghi senatori, l'atto in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ha per oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte degli studenti e dei loro familiari. Il provvedimento intende porre un argine alla successione di gravi episodi che hanno visto docenti vittime di violenza, hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona. Questa proposta di legge, a firma del collega onorevole Rossano Sasso, fortemente voluta dal Gruppo Lega-Salvini *premier* insieme agli alleati del centrodestra, interviene su due piani: da una parte, introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico; dall'altra parte, interviene sotto il profilo penalistico sanzionatorio. Prima di passare a una rapida disamina del contenuto dei sette articoli di cui è composto il provvedimento, ci tengo a dire che sono certo che questa legge non rappresenti in nessuna misura una deriva securitaria, come purtroppo ho sentito dire da qualcuno. Le uniche finalità sono volte a rinsaldare il patto scuola-famiglia e di tutelare la sicurezza degli insegnanti, restituendo loro l'autorevolezza che meritano. Auspico sul punto che in quest'Aula si possa trovare la massima convergenza. L'articolo 1 prevede l'istituzione con decreto interministeriale dell'osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, di cui fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle organizzazioni studentesche e dei genitori maggiormente rappresentativi a livello nazionale, e anche un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'osservatorio sono attribuite funzioni di monitoraggio e l'analisi delle segnalazioni di casi di violenza nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o di minaccia a danno del personale scolastico. Sono inoltre attribuite dall'osservatorio le funzioni propositive di buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico, finalizzate a prevenire e contrastare il disagio giovanile nonché anche a favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie. L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro e del personale scolastico. L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, che si celebrerà il 15 dicembre di ogni anno. La Giornata è dedicata a sensibilizzare la popolazione mediante iniziative di promozione di una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. L'articolo 4, mediante modificazione dell'articolo 61 del codice penale («Circostanze aggravanti comuni»), introduce un'ulteriore circostanza aggravante del reato, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni. L'articolo 5 interviene sull'articolo 336 del codice penale («Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale»), ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d'ufficio o del servizio. Con la novella proposta si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. L'articolo 6 modifica l'articolo 341-*bis* del codice penale («Oltraggio a pubblico ufficiale»), il quale prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Con la disposizione in commento qui si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola. L'articolo 7, invece, reca la clausola di invarianza finanziaria. Questa la sintesi. Grazie Presidente, grazie colleghi.

di quello che sta succedendo in alcune Regioni d'Italia a causa del maltempo, in modo particolare nella mia città e nella mia provincia, Vicenza, dove hanno chiuso le scuole hanno chiuso tutti i luoghi importanti di fruizione, anche della mobilità, perché in due giorni è arrivata una pioggia talmente forte, causata da forti raffiche di vento, da provocare già in molti casi l'esondazione dei fiumi Retrone e Bacchiglione in alcune parti della Provincia e anche in città. Ancora una volta, quarantotto ore quello che normalmente dovrebbe piovere in un'intera stagione invernale. C'è molta allerta e apprensione. Volevo portarvi a conoscenza di questo fenomeno, chiedendo ancora una volta al Governo che si faccia partecipe e che sia vicino a queste comunità, che, come al solito, non aspettano l'aiuto dello Stato, ma, essendo una Regione e una Provincia sempre molto laboriose, stanno incessantemente lavorando, grazie a un lavoro di squadra tra amministrazione comunale e provinciale, agli operatori, alla Protezione civile e alle Forze dell'ordine, ma anche a tutte le categorie economiche, oltre che ai cittadini, che stanno vedendo la piena, come è accaduto anche questa notte. Ancora una volta è emergenza maltempo e ancora una volta, chiedo al Governo di investire in politiche di prevenzione sulla sicurezza ambientale. *(Applausi)*. Se non diamo anche più risorse ai nostri amministratori, come facciamo a mantenere gli argini dei fiumi puliti? Tanto lavoro è stato fatto in questi anni, grazie anche all'intervento della Regione Veneto, in collaborazione con la Provincia e il Comune, per mettere in sicurezza molte parti della città e della provincia. Concludo, signora Presidente, chiedendo di non lasciare sole queste comunità, che non sono abituate a lamentarsi, che stanno lavorando e stanno dando il massimo, ininterrottamente. Noi, però, dobbiamo essere al loro fianco, come parlamentari del territorio, e con le colleghe e le colleghe e i colleghi della nostra Provincia lavoriamo sempre insieme per il nostro territorio. Quindi, vi ringrazio di avermi dato l'opportunità di intervenire anche su questo momento importante, difficile e critico che sta vivendo la città di Vicenza e tutta la provincia.

dovrebbe essere all'attenzione del Parlamento.

a volte sembrano quasi imprevedibili, in stagioni non prevedibili, ma ormai l'imprevisto sta diventando ordinario. Per fortuna, sono già stati fatti notevoli interventi. È stata lungimirante la Regione Veneto che ha lavorato sui bacini

questi fenomeni meteorologici, che si stanno verificando in maniera sempre estrema, hanno dimostrato che queste opere sono importanti. Qualcuno diceva che c'è una dittatura idraulica: l'acqua è dittatrice, l'acqua è domina

ma soprattutto un ringraziamento va a tutti coloro che si stanno adoperando, alla Protezione civile, alla Polizia locale, ai Vigili del fuoco, alla prefettura e a tutti gli organi che stanno adesso intervenendo.

Sono in contatto da ieri con i rappresentanti istituzionali della città di Vicenza, in modo particolare con il sindaco Giacomo Possamai, che sta seguendo questa situazione assai delicata, che ha portato ad in queste ore, per tentare di proteggere la popolazione, gli studenti, la città, l'intera provincia, e per garantire che non ci siano ulteriori devastazioni e danni ad una realtà importante come quella di Vicenza. Credo anch'io che sia necessario, da parte del Governo, prestare la massima attenzione a quello che sta avvenendo, per garantire tutto l'aiuto possibile alla città di Vicenza e alla Regione Veneto, perché gli interventi che dovranno essere fatti siano efficaci e realizzati in tempi veloci. Credo anch'io che in quest'Aula tutti quanti dobbiamo renderci conto

delle forze politiche del Parlamento. Questo per fare una serie di interventi che ci permettano di affrontare fenomeni come quelli che abbiamo visto in Veneto nel corso di questi mesi che hanno avuto a che fare con la siccità, per affrontare elementi e fenomeni come quelli con cui abbiamo avuto a che fare nel corso di questi anni e in questi giorni e che sono legati ad eventi atmosferici eccezionali che rischiano quindi di creare danni alla nostra realtà. È già avvenuto in altre aree del Veneto nei mesi passati; ancora non sono stati fatti tutti gli interventi necessari. Io credo che a partire da questa vicenda che riguarda la città di Vicenza sia necessario intervenire efficacemente, sostenere quel territorio con gli aiuti necessari e soprattutto fare in modo che nell'agenda culturale e politica del Governo e del Parlamento il fenomeno dei cambiamenti climatici non solo non venga negato, ma venga affrontato con la dovuta attenzione.

detto anche il collega che mi ha preceduto, questi eventi non sono più eccezionali, ma sono ormai all'ordine del giorno; pertanto, a livello parlamentare ma anche governativo, vanno accelerate tutte le

dare una *governance* che permetta di gestire questi eventi. Non possiamo reagire quando ormai sono già avvenuti, perché causano danni economici stratosferici, ma anche

di transizione energetica ed ecologica per evitare questi danni enormi, ma anche per assicurare un futuro alle nostre generazioni.

sulla questione dei fiumi: per fare una pulizia di un torrente, l'amministrazione comunale si deve rivolgere prima al Genio civile, poi magari alla Regione, poi successivamente alle Autorità di bacino. Dovremmo quindi individuare un riferimento certo che possa essere quello che deve controllare, sorvegliare e poi autorizzare la pulizia dei torrenti. Non è vero che servono soldi da dare alle amministrazioni, perché con i soldi soltanto non si risolve il problema. I soldi invece si possono incamerare incamerare dalla pulizia dei torrenti, perché basterebbe solo mettere in commercio gli inerti in eccesso che ci sono all'interno dei torrenti, anziché andare ad autorizzare delle cave a monte dei torrenti, che poi sono quelle che permettono il dilavamento del materiale alluvionale nei torrenti, e con il ricavato di quei fondi si potrebbe intervenire per ripristinare gli argini, per ripristinare le briglie, per mettere in sicurezza le sezioni e riportare la sezione originale del fosso del torrente e quindi consentire all'acqua il suo deflusso naturale. Penso che questa sia una buona occasione per cercare di lavorare insieme, con la speranza di prevenire, anziché poi dover tornare in Aula a lamentarci e magari a sostenere e dare solidarietà ai popoli che vengono purtroppo interessati da questi eventi alluvionali.

all'attenzione della Commissione competente ci sono diversi disegni di legge importanti sul consumo di suolo e mi pare che gli interventi di oggi ci possano dare qualche rassicurazione sul fatto che si possa andare avanti con questa discussione e con interventi importanti.

asterremo, perché in linea di principio siamo sicuramente d'accordo su qualunque intervento si faccia nei confronti della scuola, però riteniamo che quello previsto nel

Siamo anche d'accordo sull'istituzione di un osservatorio che possa monitorare tutte le situazioni di disagio e di violenza nelle scuole,

in Commissione sia la senatrice Bucalo sia la sottosegretaria Frassinetti - questo non può essere l'unico elemento per intervenire sulle problematiche della scuola, come il disagio giovanile o la dispersione scolastica.

e sicurezza, per migliorare l'atteggiamento dei ragazzi e delle famiglie e per incidere nella società, cosa serve? Non servono chiacchiere e distintivo,

professionisti che possano aiutare i docenti, come gli educatori, i pedagogisti, gli psicologi. Noi quindi siamo d'accordo su questo provvedimento, che è un'enunciazione di buoni intenti. E i buoni intenti per la scuola, come sa chi la conosce -

Mi metto nei panni delle figure che comporranno l'osservatorio sulla violenza, perché dovranno promuovere le buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, combattere la dispersione scolastica, il bullismo, la violenza, il disagio giovanile. E come faranno, se

Questi sono numeri che potete prendere dal sito del Ministero. Non mi sto inventando nulla. Poi c'è un altro bellissimo intento: promuovere lo svolgimento di corsi di formazione. Sono d'accordo, siamo d'accordo. Sapete quanto il ministro Valditara ha stanziato nel 2024 per la formazione docenti? Zero euro. Noi avevamo stanziato 4 milioni di euro per la formazione del corpo docente. Perché in questo provvedimento scrivete cose che avete definanziato? Perché? Lo chiedo alla Sottosegretaria, mentre i Ministri volano alti, spesso non sanno come funziona la scuola. Ma chi la scuola conosce deve sapere che, per dare dignità ai docenti, servono i soldi, servono le risorse che avete tolto. E voi invece finanziate la piattaforma! a parlare di un intervento che abbiamo sposato in maniera trasversale - lo ricordo ai colleghi della Lega - ossia l'istituzione dell'educazione civica, con tutti i limiti che porta, perché è trasversale e va migliorata. Cosa abbiamo fatto quando eravamo al Governo? Abbiamo aggiunto un piano sistemico: si chiamava piano RiGenerazione scuola. Abbiamo stanziato risorse per dare strumenti e professionisti alla scuola, per effettuare azioni di educazione civica, per lavorare sui ragazzi e con i ragazzi. Sapete quanto ha stanziato Valditara per l'educazione civica? 300.000 euro, cioè 7 euro a scuola. Come si fa? *(Applausi)*. Andate a inasprire le pene, ma cosa risolvete? La scuola ha bisogno di attenzione vera.

e alla scuola zero, 7 euro per l'educazione civica. *(Applausi)*. Che senso ha, quindi, inasprire le pene? Non lavoriamo veramente per il tessuto giovanile, per i ragazzi, per la società. Voi comunque con i numeri siete bravi, e non nella legge di bilancio, quando si tratta di stanziare soldi sulla scuola, ma per introdurre i numeri nella valutazione per i ragazzini: volete reintrodurre un numero per valutare un bambino di sette, otto, nove anni. Un numero? Un bambino di sette anni tornerà da scuola dicendo: «Ho preso 6, 7 o 10»? No, signori, ci vuole il giudizio.

E poi l'osservatorio - benissimo - è composto anche da diversi rappresentanti dei Ministeri. È bene lavorare su più fronti, ma allora pensateci bene quando strutturate altre misure. a Te, che è un'elemosina di Stato: 300 euro per chi ha necessità. Con quella carta, signori, a differenza del reddito di cittadinanza, le famiglie non possono comprare neanche un libro. Come si combatte la povertà educativa? *(Applausi)*. Neanche un libro possono comprare e con quella carta non si può comprare neanche un gioco, che spesso vale più di un pezzo di pane per un bambino e la sua formazione. Non avete visione di scuola e avete una triste visione di Paese, che sconquassa quella che è la rete sociale della nostra bella Italia che ancora sta in piedi, nonostante voi. voi. Soltanto in una cosa secondo me, per suo tramite, Presidente, sono bravissimi: sono la più importante fabbrica di *fake news* e di disinformazione della politica. Arrivo al dunque: abbiamo stanziato, con il Governo Conte II, 10 miliardi, per la scuola. Ma il mantra di questa maggioranza è sempre stato uno e lo ripeto: uno e lo ripeto: banchi a rotelle, banchi a rotelle, banchi a rotelle. Diciamo, tra parentesi, che noi abbiamo stanziato 460 milioni per gli arredi scolastici e voi in tutto il 2023, Sottosegretaria, avete stanziato 180 milioni per tutta la scuola. *(Applausi)*.

cui esiste violenza nei due luoghi laicamente sacri, la scuola

se gli alunni sentissero la violenza verbale e gli attacchi incredibilmente portati avanti in quest'Aula, che cosa ne trarrebbero? Anche nell'Aula del Senato, la Camera alta, si esercitano violenze verbali, aggressività Signor Presidente, tramite lei, dico che l'esempio parte da qua. Io sono circa cinquant'anni che mi occupo di bambini e ho sempre detto che il primo elemento pedagogicamente positivo è l'esempio. Ma che esempio diamo quando attacchiamo con questa sconcezza, questo voyerismo della maleducazione? Me lo chiedo e credo che il mio intervento sia questo. Ho sempre rispettato gli avversari; anzi, ho sempre creduto che proprio tra gli avversari, con tutto il rispetto per quello che si crede e credo profondamente, c'è democrazia. L'inconsulto attacco su tutto è veramente vergognoso. Signora Presidente, se ne faccia carico. Per quello che riguarda

al di là di provvedimenti ottimi come quello oggi in discussione, c'è da interrogarsi su che periodo stiamo vivendo e non da oggi. È troppo facile dire che è colpa loro, perché hanno il cerino in mano. mano. Io dico che certi momenti critici hanno un'evoluzione temporale di qualche anno. Tutti ci dobbiamo assumere la responsabilità. Certo, un po' meno chi, come noi, è stato tanto spesso all'opposizione.

di come si concepiscono la politica e la democrazia. A me sembra che proprio oggi stiamo facendo lo stesso gioco brutto, quello di dare la colpa a chi non c'era

Certo, non possiamo essere indifferenti alle violenze che avvengono a scuola intanto perché è veramente ingiusto, anche a livello culturale, ammettere che un insegnante debba vivere con il timore di essere - lo dico tra virgolette - a livello psicologico e addirittura fisico. Fuori i mercanti dal tempio.

non si può essere scuola-centrici: bisogna essere rispettosi di tutto l'ambiente di vita del bambino e dell'adolescente, che si vedono privare di spazi fuori dalla scuola. Bisogna ricostruire la mentalità degli oratori e degli spazi verdi, la realtà comunitaria intra ed extra scolastica. Bisogna aiutare i genitori, i politici locali e gli insegnanti a far sì che si crei una comunità che sia un tutt'uno. I pianeti girano intorno al sole: il sole è il bambino. Bisogna girare intorno a lui con rispetto, tranquillità e - diciamocela tutta - con generosità intellettuale, che stamattina non vedo in quest'Aula. Ciò mi amareggia molto

Si cerca con un'osservazione, che non significa un telescopio di qua che crea distanza, ma pur la partecipazione di quello che accade. Questo vuol dire osservare, significa interagire. Ma meno male! luogo, si costituisce la giornata che ricorda quello che dobbiamo fare. Si parla tanto di ricordi; una volta che si istituisce una giornata per pensare e ricordare, ci sembra una fetecchia. Ma, ragazzi, cerchiamo di essere leali. Il gioco è uno e non si possono cambiare le regole in corso di gioco, a seconda di quando ci fa comodo. Vorrei concludere così, però. Esistono persone protagoniste di violenza, frutto del disagio, frutto dell'ignoranza, frutto della maleducazione e del disagio mentale. Certamente c'è anche il deterrente punizione, ci mancherebbe altro. Però io credo che la cosa più importante sia quella di sentirci tutti in un gioco meraviglioso, che si chiama crescita dolce e rispettosa del bambino.

che in quest'Aula, oggi e qui, parlando del diritto di chi insegna ad avere tranquillità, si parli di manganellate. Ma che schifezza è? Ma che disturbo intellettuale c'è dietro questo? Io me lo chiedo, perché non possiamo fare i grilli parlanti qua - anche perché il grillo parlante non ha fatto una bella fine e mi dispiace - qui qui seminare zizzania e fuori dolcezza. Il doppiopesismo non c'è, soprattutto qua dentro. Grazie, Presidente, e mi scuso di aver esagerato.

prima di entrare nel merito del provvedimento, vorrei dire, a nome del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, che questa proposta di legge, questa iniziativa legislativa sicuramente ha ha il merito di intervenire su un problema - come è stato sollevato poco fa dal collega Guidi - sul tema delle aggressioni, della violenza dell'incitamento all'odio, che purtroppo abbiamo visto in molti fatti di cronaca proprio nei confronti dei docenti, sia da parte dei genitori che degli studenti.

ad una serie di violenze e di aggressioni nei confronti dei docenti, a cui vanno la nostra solidarietà e il nostro sostegno. Sono persone che molto spesso devono supplire alle mancanze familiari, a famiglie che spesso sono monogenitoriali o hanno problemi drammatici

intervenendo sull'altro provvedimento che riguardava le politiche di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Mi rivolgo al Governo e alla Sottosegretaria, che so essere molto sensibile su questi temi; spesso ne abbiamo parlato insieme, anche nella scorsa legislatura. Certamente abbiamo bisogno di investire in maniera strutturale sui temi della prevenzione e su un nuovo patto educativo tra famiglia e scuola *(Applausi)*. È chiaro che con questa proposta di legge non possiamo pensare di risolvere un problema che ci portiamo

che andava nella direzione di costruire una riforma vera del *welfare* della scuola, mettendo al centro il tema degli insegnanti, che sono sottopagati, che fanno un lavoro difficilissimo. Contemporaneamente, però, si accoglievano le richieste giuste riguardanti tantissime, migliaia di famiglie, quale quella sulla povertà educativa, la povertà digitale. C'è una generazione che ha bisogno di aiuto, che ha bisogno di essere guidata anche rispetto al tema dei *social*, al tema difficilissimo di quello che succede su Internet, tema ancora non

a fornire aiuti e sostegni reali alle famiglie, ai ragazzi, investendo in cultura, investendo in nuovi luoghi di aggregazione. Abbiamo parlato anche di sport come ulteriore strumento efficace nel contrasto a tanti problemi riguardanti le dipendenze dei nostri ragazzi. Io spero che, prima o poi, si possa aprire un dibattito serio sulle nuove droghe e anche sul ritorno dell'eroina, soprattutto nelle città più ricche, che sta distruggendo una parte importante di ragazzi, spesso minorenni. È chiaro che dobbiamo pensare che un nuovo patto educativo tra famiglia e scuola preveda, prima di tutto, investimenti strutturali. Da questo punto di vista,

di un Gruppo che crede nelle riforme, che è un partito riformista e che sta lavorando per dare anche un aiuto, un sostegno, allo stesso Governo quando ci sono situazioni su cui possiamo lavorare assieme. Quindi, da una parte, va certamente bene l'istituzione

per aiutare e prevenire fenomeni di violenza e di aggressione nei confronti del personale scolastico? C'è un tema legato all'educazione che - mi permetto di dire - è prima di tutto l'educazione ai genitori, alle famiglie. A partire dalla mia generazione, noi non ci dobbiamo sottrarre e fare anche un *mea culpa*. Il senatore Guidi parlava, giustamente, di maleducazione e la vediamo anche nei luoghi dello sport, dove spesso i genitori intervengono in maniera violenta

perché bisogna ricreare un sistema educativo, recuperare il concetto di comunità rispetto ai pilastri della nostra società, che sono questi. Penso al rispetto dei valori essenziali che ci insegnano

di relazione, di affettività, dove si formano i nostri giovani, i nostri bambini. Anche su questo dobbiamo capire cosa quali cause poi hanno portato anche all'aumento delle violenze e delle aggressioni nei confronti del personale scolastico. È quindi chiaro che serve anche un nuovo patto generazionale per intervenire in maniera efficace. Parlare di prevenzione e di contrasto alle dipendenze significa che scuola e famiglia devono investire nella comunità risorse anche in termini di personale, di formazione adeguata,

i fondi che erano stati inseriti proprio per aiutare il terzo settore e le famiglie ad avere degli aiuti. Se queste problematiche non le capiamo alla radice, è evidente che esplodono anche in fenomeni di violenza e di aggressione nei confronti del personale anche attraverso le *baby gang* che sono in aumento nelle nostre città e nei piccoli paesi. È quindi evidente che dobbiamo ricostruire una riforma del *welfare* che tenga conto di tutti questi aspetti. Bisogna fare una fotografia reale del nostro Paese che oggi è a macchia di leopardo, perché ci sono intere comunità che non hanno servizi, né strutture. Come facciamo ad aiutare

non mancheranno il nostro impegno e il nostro sostegno quando si parlerà di aiutare le famiglie, gli studenti, il personale scolastico. Però, per favore, se non costruiamo e non investiamo in politiche di lungo percorso, con una visione per i prossimi dieci anni, i pilastri fondamentali del *welfare* non andranno nella direzione

così come anche l'*escalation* dei discorsi d'odio nei confronti di chi ricopre ruoli pubblici. Esiste ormai una vera e propria diffusione sociale della violenza - la potremmo definire così che è anche il segno di una sempre più scarsa considerazione, purtroppo, del ruolo dell'insegnante, del docente e in generale della istituzione scolastica. A mio avviso, questa è una questione serissima che ha anche a che fare con un dato: la scuola italiana ha avuto per decenni un valore sociale e culturale importante, importantissimo, che però nel tempo si è profondamente smarrito. Ciò è accaduto anche perché oggi la professione di insegnante non è adeguatamente retribuita e i rinnovi contrattuali vanno troppo a rilento. Io mi aspetto davvero che dinanzi a questioni così serie il Parlamento possa fare una riflessione concreta, autentica, per ridare alla scuola pubblica quella centralità che faticosamente ha contribuito a costruire la democrazia del nostro Paese. Il mondo della scuola - a mio avviso - non crede che una stretta securitaria, cioè un mero intervento sul sistema penale, penale, possa risolvere di per sé la situazione, ma chiede che venga posta attenzione al tema grande della comunità educante. Tra l'altro, ricordo che siamo cofirmatari di un disegno di legge proprio su tale questione, che consideriamo serissima, che consideriamo serissima, perché riteniamo decisivo il tema dell'educazione delle ragazze e dei ragazzi, in particolare quello dell'educazione alla gestione delle emozioni e anche quello della formazione del personale docente. dovrebbe essere accompagnato da una formazione specifica che riguardi, per esempio, la gestione dei gruppi adolescenziali come spesso è una classe. Il Parlamento, invece, a questa proposta che sostanzialmente ne ricalca una già approvata nel 2020 e che, in quel caso, riguardava le aggressioni al personale sanitario e sociosanitario. Dico che questa proposta la ricalca perché quella legge, in sostanza, prevedeva l'istituzione di un osservatorio e anche in quel caso l'aggravamento delle pene comminate a chi si rendeva o si rende protagonista di atti di violenza contro il personale sanitario, come purtroppo - lo sappiamo bene - avviene quotidianamente negli ospedali e nei presidi sanitari italiani, al Sud Italia in particolare, purtroppo, ma non soltanto in quelle realtà. Quella legge prevedeva anche alcune norme norme riguardanti la prevenzione e quindi l'obbligo anche delle ASL di lavorare su questo punto con misure specifiche, provando a mettere in campo elementi di contrasto capaci di agire non semplicemente dopo che il fatto si era compiuto, ma anche in maniera preventiva. Pensando al provvedimento che approviamo oggi, che riguarda il mondo della scuola, se andiamo a vedere i dati che riguardano le aggressioni del personale sanitario, per verificare cioè se norme di questo tipo, che aggravano le pene, abbiano effettivamente un'efficacia oppure se non siano semplicemente azioni di propaganda, rileviamo che dal 2016 al 2020 il numero delle aggressioni al personale sanitario è rimasto, nonostante l'aggravamento delle pene, sempre costante. È sceso soltanto nel 2020, ma banalmente perché c'era la pandemia. Il *trend* degli eventi, quindi, è sostanzialmente sempre uguale. La deflessione media del 30 per cento ha riguardato, per l'appunto, soltanto l'anno della pandemia e per il resto si può dire chiaramente che quell'intervento, la scelta cioè di intervenire semplicemente sul terreno penale, non ha portato a nessun risultato. Lo stesso osservatorio ci dice che quindi non c'è stato nessun cambiamento reale nel numero degli eventi che si verificano e nemmeno nella loro qualità. L'osservatorio che queste misure non servono a granché se non sono perlomeno accompagnate da un lavoro di fondo, che poi è quello che è mancato, purtroppo, in tutti questi anni e che manca ancora: un lavoro sociale, culturale, di educazione, di formazione, che andrebbe fatto naturalmente anche e soprattutto utilizzando professionisti, figure professionali specializzate come, per esempio, quelle degli educatori, che peraltro speriamo possano essere riconosciuti attraverso l'istituzione di un albo (un disegno di legge dovrà essere approvato a breve in seconda lettura e sarebbe ovviamente una cosa significativa). È un peccato, dunque, che una misura reale di contrasto e di prevenzione delle aggressioni contro il personale scolastico, proprio perché deve avere queste caratteristiche di ricostruzione dei nessi educativi e culturali della comunità educante e delle famiglie, avrebbe però necessità di risorse e invece anche le norme che approviamo oggi

non si investe nemmeno un centesimo nel tentativo di far funzionare quelle logiche preventive che invece tanto servirebbero. Capite bene che noi consideriamo questo provvedimento che oggi approverete con la nostra astensione come una disciplina che rischia di essere molto poco significativa se non del tutto irrilevante. Noi ci asteniamo, perché all'interno di essa c'è una sola previsione dal nostro punto di vista positiva ed interessante, che è quella della istituzione di un osservatorio che segua i casi di violenza nelle scuole. Ci teniamo a sottolinearlo perché è bene che ci sia un luogo in cui venga monitorata la situazione, ma è anche importante che questo osservatorio possa avanzare proposteper abbandonare l'approccio ideologico, securitario e panpenalista per arrivare invece a un approccio di senso che possa, questo sì, davvero incidere sulla condizione degli insegnanti e delle insegnanti. In conclusione, credo

da troppe riforme, una più sbagliata dell'altra - fatemelo dire così - e da logiche aziendalistiche e finanziamenti del tutto insufficienti. Penso che la scuola abbia bisogno di risorse e di attenzione, ma che non abbia certo bisogno, signora Sottosegretaria, dei 5 in condotta e del ritorno dei voti numerici,

per ridare alla scuola la centralità che meriterebbe e che invece, questo sì, servirebbe molto per costruire un nuovo e serio patto educativo.

consentitemi innanzi tutto di esprimere vicinanza da parte del Gruppo Forza Italia alle popolazioni colpite dal maltempo degli ultimi giorni, anche ai sindaci dei Comuni interessati da questi eventi alluvionali e soprattutto al Comune di Vicenza. Oggi mi piace intervenire su questo tema non solo come senatore di Forza Italia, ma come membro di una comunità che sta vivendo un momento di profonda riflessione. Stiamo discutendo di un disegno di legge volto a proteggere il personale scolastico da atti di violenza, che testimonia la volontà di costruire una scuola più sicura e rispettosa. Tale scelta punta a ristabilire un principio fondamentale nel contesto educativo: il rispetto dell'integrità fisica e morale di coloro che dedicano la loro vita all'istruzione. Questo provvedimento non nasce, come ho sentito dire da qualcuno, da un desiderio di punizione, ma dalla necessità di proteggere e difendere la sacralità dell'ambiente scolastico, nonché di assicurare che la scuola rimanga un luogo di crescita, formazione e sicurezza per tutti. È un segnale chiaro che lo Stato non tollera violazioni contro chi ha il compito di educare e formare le future generazioni, ma al tempo stesso è un invito a riflettere sulle cause profonde che portano a tali gesti, sulla necessità di un dialogo aperto e costruttivo, sul ruolo fondamentale dell'educazione familiare e sulla responsabilità collettiva nel promuovere una cultura di rispetto e confronto civile. Non possiamo ignorare che proprio in questi giorni le nostre strade sono state teatro di manifestazioni giovanili che purtroppo hanno visto episodi di violenza

Il nostro dovere come rappresentanti delle istituzioni è di ascoltare e cercare di capire le ragioni profonde che spingono i giovani a scendere in piazza, a volte anche esprimendo i loro dissensi in modi che non possiamo condividere, ma certamente non portando qui in quest'Aula esempi di attacchi inconsulti e violenze verbali, dividendoci anche su questi temi che sono così importanti. La violenza, sia essa nelle scuole o nelle piazze, è sempre da condannare, in qualunque modo e da chiunque provenga, però è il segnale che forse non stiamo ascoltando abbastanza e stiamo trascurando le esigenze di dialogo, inclusione e comprensione che sono fondamentali per ogni società che si voglia definire matura e democratica. E non risolviamo certo la situazione

promuovere anche il fatto che ci sono 3,8 miliardi (un miliardo in più rispetto ai piani precedenti per il periodo 2021-2027) che uniscono i Fondi strutturali con quelli del PNRR, caso non è solo una questione di risorse. È qui che il nostro disegno di legge incontra la strada. Entrambi parlano della necessità di costruire ponti, di educare al rispetto reciproco, di riconoscere l'importanza del dialogo come strumento privilegiato per risolvere i conflitti. La scuola è il primo luogo dove impariamo il significato di comunità, dove sperimentiamo il confronto e l'apprendimento reciproco. È lì, proprio nella scuola, che possiamo insegnare ai giovani che ogni azione ha delle conseguenze, che il rispetto è alla base di ogni relazione civile, che il dialogo è sempre preferibile al confronto. Ma questo insegnamento non può fermarsi alle porte della scuola; deve estendersi alle nostre case, alle nostre piazze, alla società intera. Dobbiamo chiederci: come possiamo aspettarci rispetto e comprensione dai giovani se non siamo i primi a dimostrare di saper ascoltare, di cercare di comprendere le loro esigenze e le loro paure, i loro sogni? Come possiamo parlare di educazione alla non violenza se non siamo capaci di garantire che le loro proteste, espressione di un dissenso legittimo in una democrazia, siano accolte con un atteggiamento aperto e non con i manganelli? Cari colleghi, il disegno di legge che abbiamo discusso e il contesto di tensione nelle nostre strade ci offrono un'occasione unica, quella di riflettere su come possiamo essere migliori educatori, migliori ascoltatori, migliori costruttori di quella società che desideriamo lasciare in eredità ai nostri giovani. Una società che non risponda alla violenza con la violenza, ma che sappia offrire spazi di dialogo, di confronto, di crescita congiunta. E mentre procediamo ricordiamoci che il nostro impegno nei confronti dei giovani non si esaurisce con l'approvazione di un disegno di legge. Esso rappresenta solo l'inizio di un cammino che dobbiamo percorrere insieme; un cammino che richiede ascolto, pazienza e soprattutto azioni concrete volte a migliorare le loro condizioni di vita, a rafforzare le opportunità di istruzione e lavoro, a garantire spazi di espressione libera e sicura. In questo momento storico i giovani hanno mostrato una capacità di mobilitazione e un desiderio di cambiamento che non possono essere ignorati. Hanno diritto a una voce nelle decisioni che riguardano il loro futuro, a politiche che corrispondano alle loro esigenze in termini di sostenibilità, equità sociale e giustizia. È nostro dovere ascoltarli, coinvolgerli e rispondere con azioni che dimostrino la nostra fiducia nella loro capacità di costruire un mondo migliore. Concludo questo intervento con un appello alla responsabilità e all'impegno condiviso. Non lasciamo che il dialogo tra generazioni si interrompa o, peggio, si trasformi in conflitto. Lavoriamo insieme per creare le condizioni affinché la scuola, la società, le istituzioni possano essere percepite dai giovani non come antagonisti, ma come alleati nella costruzione di un futuro di pace, prosperità e armonia. Con questo voto Forza Italia si impegna a sostenere non solo la tutela del personale scolastico, ma anche l'importanza di lavorare alla radice del problema, incentivando politiche sociali, educative e familiari che possano prevenire la violenza prima che essa si manifesti. Questo dovrebbe essere un momento di unità - ho visto che molti si sono allontanati dall'Aula - un momento in cui, al di là delle appartenenze politiche, ci troviamo concordi nell'affermare che la violenza, sotto qualsiasi forma, non può e non deve trovare spazio nella nostra società e soprattutto nelle nostre scuole. Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia a questo disegno di legge, con la speranza che possa rappresentare un passo in avanti verso una scuola più sicura, più giusta e più inclusiva, ma anche verso un futuro in cui l'educazione e il rispetto siano i pilastri su cui costruire la nostra comunità.

le difficili condizioni in cui da tempo è chiamato a operare tutto il personale scolastico sono ormai sotto gli occhi di tutti. Sono felice che proprio in quest'Aula oggi siamo chiamati a riflettere su un tema così importante per tutta la comunità educante, nei confronti della quale si è leso non solo il concetto dell'autorevolezza professionale propria dell'insegnante, ma anche il principio stesso del rispetto per la persona. persona. Fuori da ogni pregiudizio, con riferimento a questo testo, è importante invitare l'Assemblea a una riflessione più attenta sulla prevenzione di ogni atto di violenza. È evidente, anche percepibile, l'esigenza di tanti docenti e operatori scolastici, che reclamano, in maniera anche molto accorata, accorata, la nostra attenzione e il nostro aiuto per consentire loro di lavorare in condizioni di sicurezza migliori. Purtroppo questo testo tocca solo marginalmente il problema. hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, in questo disegno di legge sono presenti modifiche ad alcuni articoli del codice penale, che rappresentano sicuramente un deterrente, ma non certamente una soluzione. Si introduce un'ulteriore circostanza aggravante del reato nei delitti commessi con violenza o minaccia in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale scolastico docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. È altrettanto utile mantenere viva l'attenzione sul problema, anche istituendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, com'è stato detto, il 15 dicembre. Tutto questo, però, spinge e invita i Governi e i Ministeri competenti, in questo caso quello dell'istruzione e del merito, anche a promuovere iniziative volte alla formazione e alla sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro e del personale scolastico. Peccato però che sono chiamati a intraprendere iniziative di questo tipo senza prevedere ulteriori stanziamenti e fondi; sono quindi dei buoni propositi, certamente molto condivisibili, ma se non adeguatamente

migliore per la comunità e i ragazzi, investendo di più nelle strutture, nelle palestre scolastiche, rivalorizzando gli oratori e i parchi.

quanto oggi sia in parte fuori controllo, perché spesso degenera in atti di violenza verso il personale scolastico. Abbiamo avviato in Commissione lunghe sessioni di audizione, dove a gran voce tutti hanno chiesto un aiuto e un'attenzione in più.

molteplici funzioni, ma di fatto soltanto di monitoraggio. Durante l'esame in Commissione ci siamo confrontati con altri colleghi e abbiamo cercato cercato di invitare ad un maggiore approfondimento, perché questa poteva essere l'opportunità di inserire nel testo la figura dello psicologo scolastico, ma in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e non più solo in alcune realtà, a seconda dei fondi stanziati dagli enti locali o dalle sensibilità dei dirigenti. Un soggetto certamente terzo, quello dello psicologo scolastico, che supporta gli studenti e le famiglie, capace di intercettare preventivamente, con adeguate competenze, quel malessere che coinvolge sempre di più gli studenti e che in molti casi - purtroppo è sotto gli occhi di tutti, la cronaca ce lo ricorda - si trasforma in atti non solo di intimidazione e di aggressione, ma di vera e propria violenza. C'era l'opportunità, in questo testo, di approfondire e incrementare le ore di educazione civica con docenti adeguatamente formati su tutte quelle norme utili a creare i futuri cittadini del domani, ragazzi più consapevoli, attenti, rispettosi più strutturati verso quel mondo gentile e rispettoso a cui tutti noi auspichiamo. Mi Mi avvio alla conclusione, Presidente, perché, per quanto il testo sia sostanzialmente ricco di buoni propositi, compie più un'opera di inasprimento di pene e di monitoraggio, ma non offre gli strumenti necessari davvero volti a raggiungere l'obiettivo che si pone poi questo disegno di legge, che è quello della prevenzione. Quindi, essendo questo molto lacunoso, seppur condivisibile, il Gruppo di Azione si asterrà. *(Applausi)*.

per cento di violenze dei genitori contro il personale scolastico. Alle superiori uno studente su tre afferma di essere stato testimone, almeno una volta nella sua intera carriera scolastica, di aggressioni nei confronti dei docenti, nel 70 per cento dei casi verbali. per cento dei ragazzi che hanno condiviso episodi violenti dice inoltre che durante lo svolgersi dei fatti qualcuno si è occupato di riprendere le scene. cento dei casi i genitori si schierano dalla parte dei figli, mentre gli insegnanti, vittime, solo nel 15 per cento dei casi segnalano quanto avvenuto alla Presidenza. Secondo altri dati forniti recentemente dalla UIL Scuola, nel 6 per cento degli istituti superiori lombardi è stato necessario ricorrere all'intervento della pubblica autorità. Questi sono alcuni dei dati del fenomeno che stiamo vivendo. È per questo motivo che, per iniziativa della Lega e, in particolare, dell'onorevole Sasso, è stato promosso il disegno di legge che oggi discutiamo e che intende aumentare le tutele e la sicurezza del personale scolastico. Esso nasce dalla convinzione che occorre intervenire con urgenza, ma anche con la consapevolezza che l'aspetto sanzionatorio debba accompagnarsi ad un più profondo lavoro culturale, come è stato giustamente ricordato a più riprese dal ministro dell'istruzione e del merito Valditara. Quello che affrontiamo non è infatti un normale fenomeno di ordine pubblico; l'aggressione ai docenti segnala un rapporto, divenuto spesso patologico, fra le famiglie e la scuola che compromette alla base quella necessaria collaborazione fra i soggetti che devono presiedere alla formazione e all'educazione dei nostri giovani. Negli ultimi anni infatti molti genitori - non tutti, ma molti hanno sempre più concepito il proprio ruolo come quello di difensori e protettori dei loro figli, vedendo negli insegnanti una controparte e non dei necessari cooperatori della crescita culturale e civile delle giovani generazioni. Alle spalle di questa idea c'è anche un retroterra culturale, affermatosi nel lungo Sessantotto italiano, teso ad eliminare, in nome di un falso concetto di democrazia o di uguaglianza, ogni principio di autorità nelle istituzioni scolastiche. Bisogna invece accettare che gli insegnanti siano severi e rigorosi quando è necessario, facendo pesare in questo modo la loro credibilità e autorevolezza. Il loro compito, come diceva Pasteur, non è quello di risparmiare ai nostri figli le difficoltà della vita, ma di insegnare loro a superarle. più generale quindi è quello del ruolo sociale dell'insegnante, tenuto sempre nella massima considerazione in ogni civiltà, ma oggi eroso e svilito da più punti di vista, compreso quello di un trattamento economico non sempre adeguato. Lavorare per la rivalutazione dell'insegnamento, come sta facendo il ministro Valditara, è necessario e vitale per le sorti stesse della nostra società e anche della nostra democrazia. Equiparare insegnanti e allievi, come fa certa cultura contemporanea, finisce infatti per far perdere di vista i fini essenziali della scuola, la trasmissione del sapere da una generazione all'altra, da una parte, e la formazione di una personalità matura in ragazzi che per la loro età ancora non l'hanno, dall'altra. Il ruolo di mediazione svolto dagli insegnanti non può certo essere depotenziato. Peggio ancora non si può permettere che attorno a loro si crei un contesto di pericolo e insicurezza costante. È necessario quindi che i docenti siano messi in condizioni di svolgere con la dovuta tranquillità il delicato compito che la società ha loro affidato. Senza rispetto reciproco, nella diversità dei ruoli e anche delle gerarchie fra allievi e docenti, così come senza la fiducia dei genitori nei confronti degli insegnanti, nessun corretto e serio rapporto educativo può essere instaurato. Per raggiungere questi fini la proposta di legge prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico che aiuti a prevenire la violenza nei loro confronti, individuando i contesti a rischio e mettendo in atto le precauzioni necessarie. Non viene dimenticata nemmeno la necessaria opera di sensibilizzazione della popolazione su queste tematiche attraverso un'opportuna informazione e comunicazione istituzionale. per suo tramite, Presidente, fare un po' di chiarezza sui numeri che sono stati fatti, in particolar modo dalla collega del Gruppo MoVimento 5 stelle. Si parlava di azzeramento della formazione per i docenti. Originariamente il fondo per la formazione dei docenti era pari a 40 milioni. Sì, è vero, è stato azzerato, ma non da questo Governo, che ha invece ripristinato il fondo a 40 milioni per i docenti in legge di bilancio ulteriori 200 milioni di fondi aggiuntivi per Agenda Sud, docente *tutor* e appunto la formazione. la collega - sempre per suo tramite, Presidente - sul fatto che noi non vogliamo, per i nostri ragazzi, né una scuola dei manganelli, né lo spreco pubblico dei banchi a rotelle. che i nostri insegnanti vengano rispettati per il loro lavoro e pagati quanto dovuto. In questo senso va l'aumento in busta paga voluto e stanziato da questo Governo per i nostri insegnanti. Questi sono fatti, non sono banchi a rotelle. Vogliamo che la nostra scuola sia sempre più vicina al mondo dell'impresa, come giustamente sta facendo il nostro Ministro, per avere dei ragazzi che quando finiscono il proprio ciclo scolastico trovino immediatamente lavoro e non diventino degli aspiranti percettori del reddito di cittadinanza. *(Applausi)*. La Lega richiama in questo senso tutte le forze politiche ad esercitare il massimo della responsabilità verso questa fondamentale battaglia di civiltà. È per questo che annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo della Lega.

di stamattina - è indifferente o sottovaluta gli episodi di violenza che si verificano all'interno delle scuole e che hanno toccato i docenti, il personale scolastico e gli studenti. Anzi, noi vogliamo dare peso e rilievo a questi episodi: sono preoccupanti, allarmanti e vanno contrastati. Essi sono la spia - lo diceva prima il senatore De Cristofaro - di una presenza sempre più diffusa della violenza nelle relazioni sociali quindi anche la spia di una desertificazione della società. Però, intervenendo a motivare il voto di astensione - lo dico subito - del Gruppo Partito Democratico su questo provvedimento,

Ma il diritto penale non è la soluzione di tutti i mali. Quando la politica si rivolge sempre e solo a questo strumento, non solo definisce una società del controllo e della disciplina, ma abdica al suo ruolo di comprensione, di prevenzione, di trasformazione e di governo dei processi. Tanto più in un luogo così strategico e delicato come la scuola, che è il luogo dell'educazione, della relazione educativa, del dialogo e della cittadinanza. Come 7a Commissione del Senato noi non avevamo aspettato questo disegno di legge per affrontare questi temi (lo ricordano bene i miei colleghi). Abbiamo avuto un ciclo di audizioni per un affare assegnato e abbiamo approvato uno schema di risoluzione articolato che indicava interventi su più fronti, per riconoscere centralità e autorevolezza alla figura dei docenti, ricomporre il patto educativo tra scuola e famiglie (perché di questo stiamo parlando), riconoscere e contrastare le situazioni di disagio sociale e culturale (perché la scuola non è un'isola, ma è dentro un contesto sociale e culturale) e i fenomeni di dispersione scolastica. In particolare, avevamo ripreso le importanti affermazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione: aggressività e violenza, di qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in particolare nella scuola, importante primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di una visione della persona e della società, del suo essere ed essere nel mondo come soggetto attivo, responsabile e solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo-educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei cittadini, che garantisce l'incontro e il confronto fra generazioni, l'elaborazione dei saperi e la trasmissione del patrimonio culturale di un popolo. Una risoluzione che parlava di rafforzamento del tempo scuola, di superamento del precariato e di interventi plurali. Spiace, pertanto, che, anche forti di un nostro percorso, arrivato questo testo approvato alla Camera non abbiamo potuto arricchirlo e modificarlo in alcun modo. Tutti i nostri emendamenti, neanche a dirlo, sono stati bocciati: emendamenti che andavano nella direzione di dare più forza a delle misure che pure in questo testo ci sono (come l'osservatorio, come l'informazione, come la giornata dedicata), ma dando più forza strumenti alla comunità educante nel suo complesso. In Commissione stiamo discutendo un disegno di legge a prima firma Malpezzi e su questo stiamo facendo le audizioni. Potevamo perciò cogliere dei suggerimenti da quel percorso, perché un reato commesso all'interno della scuola ha un rilievo maggiore, richiede interventi preventivi più intensi e significativi, perché il disagio che gli atti di violenza segnalano richiede una strategia che chiama in causa la comunità nel suo complesso. Quello che avviene nella scuola riguarda la società nel suo complesso. Prima delle norme penali, quindi, dovremmo leggere il carico di malessere e di sofferenza che viene registrato da diversi anni, aumentato dall'emergenza sanitaria del Covid-19, che ha segnato il mondo della scuola e le relazioni tra le persone. Ce lo dicono i ragazzi quando chiedono lo psicologo, una grande richiesta di questa generazione, e quando lamentano il malessere che vivono. Questa complessità Questa complessità noi abbiamo cercato di inserire nell'Osservatorio e di inserire nella comunità educante, prevedendo il ricorso a figure di sostegno quali educatori, pedagogisti, psicologi. Di questa complessità, nulla è stato colto. Rimangono le riforme del codice penale, rimane un osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico, rimane una giornata dedicata, ma tutto a invarianza finanziaria. Qui diventa evidente che l'unica cosa che resta del testo è l'intervento sul codice penale. Perché quale azione si può promuovere senza risorse adeguate? Anzi, semplicemente senza risorse? Dunque, ancora una volta, prevedete una norma penale, uno *spot*, forse a beneficio della stampa, che cerca di rassicurare qualche docente, ma non si vede nessuna politica che provi davvero a evitare che i fenomeni di violenza si verifichino, a prevenirli realmente, a riconoscere ai docenti la loro professionalità e autorevolezza. La La trappola dell'abuso del diritto penale è proprio questa: trasformando tutti i docenti in vittime, paradossalmente se ne cancella il ruolo attivo di trasformazione delle relazioni nella scuola, di agenti di cambiamento, di educatori. Per questo è sbagliato intervenire solo su questo versante. Ma non servirebbe neanche l'unico che conoscete, dal decreto Caivano al decreto rave: punire e punire, ossessione che rischia di criminalizzare un'intera generazione. Ascolteremo attentamente giovedì il ministro Piantedosi, perché siamo ancora impressionati dalle dalle immagini di Pisa e di Firenze. *(Applausi)*. Qui, però, siamo dentro la scuola. Restano ferme le responsabilità penali e la necessità di sanzionare i colpevoli. Ma ciò non serve e non basta, se non si affrontano i nodi strutturali, se non si ricostruisce l'alleanza tra scuola e famiglia, se non si restituisce alla scuola la sua funzione di istituzione fondante della più ampia comunità democratica e non di un servizio a risposta per interessi soggettivi. è la grande questione che ci hanno posto i sindacati nelle loro audizioni in Commissione: la scuola non è un servizio a risposta individuale. Lo stesso terribile errore state compiendo sulla valutazione. Volete cancellare il giudizio descrittivo nella scuola primaria. Ripensateci, ascoltate il mondo della scuola. La strada, in questo ed in quel caso, è rafforzare la relazione educativa, il senso del fare scuola, che non è solo la funzione selettiva e sanzionatoria, ma è l'opportunità di promozione umana nella sua complessità, restituendo centralità alla scuola pubblica. Dichiaro per questi motivi, per l'inadeguatezza di questo testo, il voto di astensione del Gruppo Partito Democratico.

altri presi di mira con pallini di gomma mentre sono in cattedra, presidi schiaffeggiati, personale scolastico aggredito da familiari degli alunni. Nel 2023 ci sono stati in tutto 36 casi; con l'aggressione avvenuta a Parma salgono già a 28 i casi di violenza e aggressione ai danni di docenti e personale scolastico dall'inizio dell'anno. È evidente a tutti che qualcosa si è rotto. La scuola ha perso la sua identità democratica e soprattutto è venuto meno il patto educativo tra la famiglia e gli insegnanti. Non si tratta di eccezioni: moltissimi colloqui con gli insegnanti finiscono spesso in discussioni accese in cui il genitore prende le parti del figlio o sminuisce la gravità degli atti gravissimi compiuti in ragazzate, fino a spingersi a comportamenti violenti contro chi da da sempre ha lo scopo di aiutare progressivamente i discenti ad apprendere, a crescere, a diventare autonomi e responsabili delle proprie scelte di vita, di lavoro e di relazione. Non è possibile che un insegnante debba costantemente avere il timore di cosa può succedergli nello svolgere il proprio lavoro, di assegnare un giudizio negativo. Il percorso di formazione è fatto di prove da superare e quelle che apparentemente sembrano le più dure e negative sono quelle che, invece, continuano a farci crescere. Non possiamo lasciare la scuola a chi lavora e si sente costantemente in una condizione di isolamento, mortificati nella loro autorevolezza e nel rispetto per la propria persona. Il provvedimento in esame interviene sostanzialmente su due piani: su quello della prevenzione, istituisce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, con l'obiettivo primario di monitorare e studiare il fenomeno e di promuovere azioni di sensibilizzazione e di contrasto; sul piano della repressione del fenomeno, interviene con una misura di natura penale, introducendo all'articolo 61 del codice nei delitti commessi con violenza e con minaccia, l'aver agito in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, e ausiliario della scuola, e all'articolo 336 del codice penale, rafforzando la natura di pubblico ufficiale del dirigente scolastico e del personale docente, introducendo un'aggravante che prevede, nel caso siano aggrediti, l'aumento della pena da un terzo a due terzi, se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore dell'alunno. Infine si istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. Presidente, oggi più che mai bisogna superare l'idea assai diffusa che la scuola non costituisca più lo strumento decisivo di crescita e di promozione personale e sociale dei nostri giovani. Senza scuola, non solo non c'è istruzione, ma non c'è coscienza sociale. Bisogna superare il dualismo che vede contrapposti da una parte la scuola e chi la rappresenta e dall'altra i genitori, in un rapporto

che rimetta al centro il destino dei nostri figli, perché la scuola non ha il solo compito di traghettare i nostri figli nel mondo della conoscenza, ma ha quello più importante di farli crescere. La scuola è il luogo per eccellenza in cui far maturare consapevolezza civica, intelligenza e rispetto delle istituzioni, condivisione dei principi e delle regole della convivenza democratica, motivazione alla partecipazione attiva alla vita della comunità, esperienze di solidarietà. È il luogo in cui i nostri figli diventano cittadini consapevoli, un ruolo che può concretizzarsi solo se alla base vi sono il confronto, la costruzione di rapporti di fiducia e lo sviluppo di una vera collaborazione tra scuola e famiglia. In caso contrario, c'è il rischio serio che le nuove generazioni saranno sempre più fragili e socialmente più divise. [**Presidenza del presidente e il ministro Valditara, oltre a conoscere bene la scuola, fin dal primo giorno hanno investito su questa grande istituzione e non con provvedimenti che di fatto hanno solo sperperato i soldi dei cittadini come hanno fatto i precedenti Governi. Alcuni esempi? Abbiamo chiuso un contratto da anni atteso da tutto il mondo della scuola, con aumenti consistenti, abbiamo approvato delle linee guide che attuano la riforma inserita nel PNRR, che prevede un investimento di 600 milioni di euro per rafforzare l'educazione e la formazione degli studenti e di 450 milioni di euro per la formazione dei docenti. Presidente, mi rivolgo alla sua persona e mi rivolgo al MoVimento 5 Stelle: tutti siamo concordi oggi nel dire no ad ogni forma di violenza è necessario, per il bene dei nostri figli, che la scuola venga custodita e difesa, quindi smettetela di strumentalizzare i nostri studenti e le loro famiglie

discutere ed approvare l'Atto Senato 931, un disegno di legge

Nonostante il rinnovato interesse per l'agricoltura, che sappiamo in questo periodo essere un settore molto attenzionato a tutti i livelli, a partire dall'Europa, per arrivare a quello nazionale, ma anche regionale e locale, che abbiamo anche testimonianza dell'attenzione di molti consumatori verso i prodotti di qualità, tipici e locali e della crescente consapevolezza in materia ambientale, l'inserimento dei giovani nel settore agricolo continua a presentare

oltre agli effetti del clima pesano sull'agricoltura italiana alcune debolezze strutturali, quali la scarsa presenza di giovani capi azienda (che si attesta solo al 9 per

del nostro Gruppo, ma credo anche di questa maggioranza, occorrono pertanto misure concrete, che permettano ai giovani non solo l'insediamento, ma anche il mantenimento e la permanenza nell'agricoltura in modo sostenibile, al fine di garantire un'attenzione concreta ai giovani in un settore strategico del nostro Paese. Il provvedimento rappresenta quindi una priorità per l'agricoltura italiana e le politiche volte a tal fine costituiscono una leva fondamentale per la ristrutturazione in termini di maggior competitività del settore primario. Le sue finalità consistono nella promozione e nel sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento, la permanenza e soprattutto un tema molto importante, ossia il ricambio generazionale.

Abbiamo poi un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani, che viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinato anche a cofinanziare a cofinanziare i provvedimenti di natura regionale o delle Province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura. Queste risorse sono volte, in modo particolare, ad agevolare l'acquisto di terreni, di strutture necessarie per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola, di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, alla manutenzione dei terreni, al processo di coltivazione dei prodotti, attraverso quelle che sono ormai definite le tecniche di precisione, l'ampliamento dell'unità minima produttiva, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, l'impiego di manodopera, l'acquisto di complessi aziendali già operativi. Si ritiene anche importante inserire un regime fiscale agevolato per il primo insediamento insediamento delle imprese giovanili, che introduce la possibilità per il giovane che intraprende questa attività di optare per un regime fiscale consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile, costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che le imprese giovanili non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività agricola e che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. L'agevolazione non deve avere a oggetto fattispecie riferibili a trasferimenti aziendali e ad altri casi. Vi sono poi le agevolazioni in materia di compravendita di fondi. Si interviene, in caso di compravendita in caso di compravendita con contratti aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore ai 200.000 euro, sul compenso per l'attività notarile, determinato nella misura prevista dalla tabella notarile vigente, ridotta della metà. vi è la possibilità di avere un credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione pari all'80 per cento, per un importo massimo di 2.500 euro. Ci sono anche agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate, con una riduzione del 60 per cento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, in favore dei giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto e iscritti, naturalmente, alla gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze. Poi abbiamo la prelazione. Voi sapete che in tema di agricoltura è determinante anche la prelazione quando si acquistano terreni confinanti. sostiene il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione tra più soggetti confinanti, prevedendo un favore nei riguardi del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo che

membri del Ministero, di Ismea, di Iccrea, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore agricolo e le associazioni dei giovani operanti nel settore agricolo e agroalimentare. C'è ancora un punto molto importante che vorrei citare, ossia la vendita diretta dei prodotti agricoli,

dobbiamo individuare nei casi negativi, ma solo ed esclusivamente nella positività del lavoro che sta facendo per garantire la filiera di un cibo sano, salubre, genuino destinato ai consumatori, non solo italiani. Ricordiamoci sempre, infatti, che quello che stiamo portando avanti il primo passo di una filiera del *made in Italy* che è straordinariamente forte. Anche quello che stanno portando avanti in questi mesi il Governo e tutte le associazioni sindacali di categoria, in risposta alle proteste degli agricoltori

sulle emissioni industriali, hanno consentito al nostro Paese un rafforzamento di queste posizioni, soprattutto in difesa degli agricoltori e dei nostri allevatori. *(Applausi)*.

oggi fa quasi sorridere, arrivando in Aula - nonostante un percorso anche abbastanza lungo, ma talvolta davvero il diavolo sembra metterci lo zampino

Giustamente gli agricoltori hanno protestato, chiedendo aiuti concreti al settore agricolo, sono seguite precipitose riunioni di Governo e, alla fine, forse sarà ripristinato.

quasi muscolare con il quale vorrebbe cercare di convincere di fare un provvedimento con il quale effettivamente si danno strumenti e, invece, come direbbero a scuola, lo studente è intelligente, ma non si applica o meglio non si applica abbastanza, alle cose ci arriva, le sfiora, è quasi all'obiettivo, ma all'ultimo momento - non so perché - non riesce a concludere, non stringe su questi provvedimenti. Dico questo perché tante cose si possono fare per il settore agricolo giovanile, ma di tutte queste cose purtroppo nel testo al nostro esame non trovo nulla. Non trovo nulla di specifico, non troviamo nulla che sia effettivamente

chi si occupava dell'agricoltura e infatti abbiamo un dato abbastanza preciso e specifico. Questo dato ci dice intanto che il settore agricolo giovanile è in crisi. Noi abbiamo sicuramente la quota di agricoltori giovani più bassa d'Europa e, tra i giovani,

di penetrazione sul mercato perché è un settore che è in mano a imprenditori grandi, a imprese soprattutto a conduzione familiare, che non sono orientate a fare entrare i giovani, a meno che non ci sia una vicenda di impresa familiare. familiare. Come al solito, con questo nostro approccio per il quale la concorrenza non ci piace, il principio di economia e di concorrenza comunitario non ci piace, anzi lo osteggiamo, invece di favorire l'ingresso e quindi cercare di superare questa barriera all'accesso, addirittura rafforziamo il patto patto di famiglia, rafforziamo sempre questo passaggio familiare e generazionale, che in sé e per sé non ha nulla di male, è ovvio. È chiaro che le tradizioni a conduzione familiare si devono difendere e tutelare; ma è l'approccio che, come sempre, è sbagliato, perché irrigidisce il mercato e non favorisce l'ingresso. Prova ne sia che appunto i giovani hanno difficoltà ad accedere. Inoltre, c'è un'ulteriore particolarità. Non soltanto i giovani hanno difficoltà ad accedere al settore perché non provengono già da esso, e quindi è difficile riuscire a trovare i terreni e le risorse per avviare un'impresa agricola, ma l'ulteriore difficoltà che hanno è sul tipo di produzione che si fa. Mi spiego meglio. Sempre il settimo censimento dice che i giovani imprenditori agricoli si differenziano dagli altri per due per due motivi: in primo luogo perché hanno un approccio multidisciplinare al settore agricolo, cioè non si limitano a coltivare, ma spesso associano alla coltivazione un agriturismo una fattoria didattica, cioè una serie di attività collaterali, che però sviluppano effettivamente anche la sensibilità agricola. Mi sarebbe piaciuto trovare in questo testo di legge qualcosa di specifico anche su questo tema; ma non c'è. La seconda cosa che ci dice sempre il censimento è che i giovani agricoltori chiaramente favoriscono le coltivazioni biologiche. È ovvio, c'è una maggiore sensibilità e quindi una maggiore volontà di portare avanti dei sistemi di coltivazione più evoluti. Anche in questo caso, in questo disegno di legge mi sarebbe piaciuto che ci fosse una misura specifica, conformemente a quelle che sono le linee di indirizzo della PAC sulla coltivazione biologica e sull'utilizzo di strumenti diversi di coltivazione. *(Applausi)*. Ma chiaramente tutto ciò in questo testo non c'è.

ma non raggiunge la sufficienza, perché gli manca sempre qualcosa. Gli manca effettivamente una visione di strumenti efficaci che davvero consentano di sviluppare e incentivare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Non bastano questi strumenti, perché il fondo perduto da 15 milioni di euro in sé e per sé in questo modo non basta. E non basta perché i sistemi di defiscalizzazione sono troppo ridotti rispetto alle esigenze. In Commissione, anche alla Camera, ci si era battuti e sembrava di aver raggiunto una condivisione di intenti con il Governo per un esonero contributivo che fosse, almeno per i primi tre anni, al 100 per cento. In tal modo si sarebbe dato veramente uno strumento per incentivare e per sviluppare questo settore. Invece dall'esonero contributivo siamo passati a una defiscalizzazione, con l'applicazione di un'aliquota al 12,5 solo per i primi tre anni, anzi per il primo anno di esercizio e per i successivi tre; quindi in totale quattro anni. Ma non a tutti: soltanto a condizione che nei precedenti tre anni dall'entrata in vigore di questa legge non si sia fatta attività imprenditoriale nel settore agricolo. Questo è paradossale,

Lo posso avere soltanto se da oggi in poi decido di dedicarmi all'agricoltura, mentre quello che ho fatto prima è come se non valesse nulla. E allora, diciamocelo, questo non è un modo per incentivare l'agricoltura; questo è un modo per dire che, da questo momento in poi, distribuiamo piccole mance per l'agricoltura, ma non vi diamo gli strumenti effettivi per farla. Non ve li diamo anche perché il credito d'imposta, quella bella misura del credito d'imposta, che si poteva dare anche per l'acquisto di macchinari e si poteva dare proprio per permettere a questi giovani imprenditori di entrare nel settore e di superare le rigidità e le barriere all'accesso,

se vogliono dare una dimensione strutturata a quella che può essere una passione? Tanti iniziano a fare tale mestiere per passione. Con quale misura questo Governo pensa di promuovere il settore agricolo giovanile? Queste sono le domande che ci facciamo e per le quali, a nome di

Signor Presidente, la discussione di questo provvedimento si inserisce in un periodo quanto mai preoccupante e drammatico per il settore agricolo, oggi al centro del dibattito politico per la protesta dei trattori che da settimane sta catalizzando l'attenzione del Paese. Alle sacrosante richieste degli agricoltori, notoriamente i soggetti più deboli nella filiera agroalimentare, che ogni giorno devono confrontarsi con gli effetti devastanti della crisi climatica e con un mercato sempre più competitivo e globalizzato, il Governo Meloni risponde, anche con questo provvedimento, in modo superficiale e deludente, introducendo strumenti fragili e inconsistenti, che in alcun modo rilanciano e sostengono il settore produttivo agricolo. Gli scontri verificatisi tra gli agricoltori e l'Esecutivo ci forniscono l'esatta sintesi del fare politico di questa destra che, lungi dall'affrontare nel concreto i veri problemi dell'Italia, continua a sfornare decreti e disegni di legge superficiali e di basso peso specifico, sottraendosi alle grandi sfide ambientali, economiche e occupazionali, che vanno colte ora e non in un futuro indefinito.

votata in sede europea da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e non da noi. Tale PAC oggi avvantaggia le multinazionali, cui è destinato circa l'80 per cento del bilancio europeo, lasciando indietro i piccoli agricoltori. Il Governo Meloni, invece, se la prende irresponsabilmente con il *Green Deal*. Non sapendo che pesci prendere, mortifica e svilisce le misure necessarie a traguardare l'obiettivo di transizione energetica ed ecologica, processo volto anche ad assicurare un futuro alla produzione agroalimentare italiana e a rendere, di riflesso, economicamente più solide anche le aziende agricole in difficoltà. La stessa identica paralizzante *ratio* sorregge anche questo provvedimento, nel quale, a fronte degli insufficienti incentivi previsti per i giovani imprenditori agricoli, sono minimamente contemplati né la dimensione ambientale né un paradigma di agricoltura innovativo e ambientalmente sostenibile. Manca una visione agroecologica che possa aiutare gli agricoltori nei vari processi di conversione ormai già in atto e traghettarli verso un'agricoltura di precisione e digitalizzata. Pensiamo solo, ad esempio, ai sistemi di irrigazione più intelligenti e precisi, con i quali gli agricoltori possono migliorare ed efficientare l'utilizzo dell'acqua, risorsa preziosa specialmente durante i periodi di siccità che si abbattono sempre più frequentemente sulla nostra penisola. Stando ai dati di Coldiretti, i fenomeni siccitosi hanno causato, nel solo 2022, sei miliardi di danni alle imprese agricole e un calo del 10 per cento della produzione agroalimentare nazionale. E, se non è siccità, sono alluvioni o allagamenti. Il provvedimento in esame istituisce, inoltre, un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, dalla cifra ridicola di 15 milioni di euro per il 2024, senza comunque subordinare l'erogazione di questi incentivi alla sussistenza dei criteri europei e nazionali di sostenibilità ambientali previsti per le imprese. Non si premiano, quindi, le *startup* più attente all'ambiente. Così, uno strumento che potrebbe costituire un importante fattore di traino, sia per l'attuazione di un ricambio generazionale nel settore agricolo sia per l'adozione di strumenti in grado di ridurre le emissioni climalteranti e razionalizzare l'utilizzo delle risorse naturali, si limita ad essere il solito presunto contentino, che però non soddisfa più nessuno. Ignorando anche la strategia Farm to Fork in tema di riconversione di sistemi agricoli e mancando di sfruttare l'opportunità di cambiamento offerta dalle nuove tecnologie, questa politica si conferma inefficiente e per niente lungimirante, deludendo le aspettative del comparto agricolo già in crisi per le politiche aziendali dettate dalla grande filiera di distribuzione. Così, tra le tipologie di interventi finanziabili in questo provvedimento ci sono l'acquisto di terreni, l'acquisto di complessi aziendali già operativi, l'acquisto di beni destinati alla coltivazione e alla manutenzione naturale dei terreni: tutte operazioni legate ad un concetto di agricoltura convenzionale oggi non più sostenibile. Utili sarebbero stati, invece, incentivi volti a diminuire l'impiego dei pesticidi, come pure noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo proposto, anche in vista del raggiungimento dell'obiettivo, fissato dalla strategia europea sulla biodiversità, di ridurre del 50 per cento l'uso dei pesticidi entro il 2031.

si colloca al sesto posto nella *top ten* mondiale per l'utilizzo di pesticidi e di altri composti chimici in agricoltura, per un totale di 114.000 tonnellate l'anno e di circa 400 sostanze diverse. Ciò vuol dire che un terzo dei cibi che ogni giorno arriva sulle nostre tavole è contaminato, quindi potenzialmente dannoso per la nostra salute. della genuinità dei cibi *made in Italy* che vi preoccupate di difendere anche attraverso ben note campagne di strumentalizzazione contro i prodotti del futuro, come la carne coltivata. È evidente che non vi rendete conto che la tutela dei nostri eccellenti prodotti tipici, che ci fanno conoscere e apprezzare in tutto il mondo, passa necessariamente anche attraverso la tutela della in tutto il mondo, passa necessariamente anche attraverso la tutela della biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente e dei nostri fragili ecosistemi. Mi spaventano molto la faciloneria e la superficialità con la quale vi approcciate ad un tema così serio come quello ambientale; argomento che interessa da vicino il futuro di tutti i settori produttivi italiani, anche quello agroalimentare, e tanto più il futuro dei giovani agricoltori che pensate di tutelare con quei ridicoli 15 milioni di euro. Lo stesso discorso vale per le altre nostre proposte emendative che non avete neanche valutato, come l'opportunità di elargire fondi ai giovani imprenditori che intendono intraprendere nuove tecniche di allevamento, anche attraverso una riduzione del numero di capi allevati. Vi ricordo che i liquami che provengono dal settore zootecnico intensivo costituiscono una delle principali cause di inquinamento dei suoli e delle falde acquifere. Inoltre, l'enorme contributo di ammoniaca che da questi deriva si trasforma in atmosfera in polveri sottili molto pericolose anche per la salute umana. Lo dico tanto per ricordarlo al ministro Lollobrigida, fortemente convinto della bontà di questi metodi di produzione convenzionali, ormai non solo dichiaratamente insostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, ma anche insufficienti a soddisfare la richiesta dei consumatori. richiesta dei consumatori. Ribadiamo che bisogna puntare sulla promozione di strumenti che consentano una riconversione dei metodi di produzione agricola in chiave sostenibile, tutelando il patrimonio idrico, preservando la biodiversità, incentivando la produzione di agricolture biologiche e sostenendo concretamente i piccoli agricoltori nella produzione, vendita e distribuzione dei propri prodotti lungo la filiera agroalimentare. In conclusione, per questo e per i motivi sopra elencati, il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra dichiara il voto contrario sul provvedimento

Presidente, ho sentito molte parole e molti ragionamenti da parte delle opposizioni a conforto di voti contrari e di astensione, tra l'altro anche in contraddizione tra loro, che quindi non troverebbero mai una vera sintesi e una direzione. Quello che dobbiamo capire è se dobbiamo e vogliamo davvero aiutare l'agricoltura e i giovani che vogliono cimentarsi con questa attività o meno, tra l'altro nel momento in cui gli agricoltori scendono in piazza in Italia, a Bruxelles, in altri Paesi europei.

con i ma, con i se, con il benaltrismo, non si va da nessuna parte, si guarda altrove senza arrivare a nessun vero obiettivo. Favorire la permanenza, ovvero l'insediamento dei giovani nelle campagne ha sia lo scopo di rilanciare il settore agricolo, sia quello di mantenere quel forte presidio del territorio che rappresenta la migliore risposta alla salvaguardia dell'ambiente, non solo nei territori montani. E va evidenziato che questo è un disegno di legge ordinamentale al quale certo devono seguire quelle risorse che - come sappiamo sono in larga parte decise dalla politica agricola comune. Ma sappiamo anche che l'agricoltura vive in larga parte grazie agli aiuti comunitari, che ovviamente sono poi alimentati dai Paesi membri, quindi dalle nostre risorse nazionali inviate a Bruxelles. Proprio in queste ore a Bruxelles viene giustamente ripensata la Politica agricola comune, con un ripensamento che vede protagonista anche il nostro Paese, nell'evidenziare quali temi e quali problemi vanno affrontati e risolti. C'è un problema evidente di rappresentanza del mondo agricolo, posto che la protesta ha portato anche con sé nuovi raggruppamenti spontanei di agricoltori, che hanno creato nuove sigle e che probabilmente erano stati dimenticati. quindi, deve trovare delle risposte concrete che devono passare attraverso una Politica agricola comune più semplice, meno legata a regole burocratiche che escludono dalle provvidenze e dagli incentivi anche alcune categorie di aziende. Va poi detto con chiarezza che l'agricoltore non può essere un ragioniere o un tecnico e, quindi, anche i meccanismi con cui si supportano le attività agricole vanno semplificati. È questione non solo di risorse da mettere, ma anche di meccanismi che devono semplificare la vita di chi vuole impegnarsi in un'attività fondamentale per il nostro Paese e la nostra Europa. Sappiamo benissimo che poche sono le attività dell'agricoltura e della zootecnia che possono dare reddito indipendentemente dai sussidi e dagli aiuti, che stanno da sole sul mercato. Sappiamo che la concorrenza che viene ai nostri agricoltori dai prodotti esteri è spietata, spesso anche sleale. E di fronte a queste sfide di Paesi senza regole non possiamo e non dobbiamo ridurre la capacità produttiva dell'agricoltura europea e italiana. Peraltro, in alcuni casi ci sono dei vincoli assurdi che all'estero non hanno e non hanno alcuna intenzione di mettere, che costringono i nostri agricoltori a rispettare determinati paletti ambientali e non, che sono dei vincoli restrittivi alle loro attività e, quindi, si ripercuotono poi anche sui risultati che noi chiediamo, ma che non possiamo avere. Le risorse sono tante, considerato che la PAC gestisce 390 miliardi, cioè circa un terzo del bilancio dell'Unione europea 2021-2027, ma bisogna bilanciarle meglio e farle arrivare a tutti, e non solo ad alcuni settori. Bisogna ridurre oneri fiscali inutili, burocrazia inutile e controlli a carico degli agricoltori che sottraggono risorse al settore. C'è poi il tema del libero scambio che avviene con Paesi extra UE che producono prodotti - come dicevo prima - senza i vincoli che abbiamo in Italia. Sono temi grandi che riguardano un settore fondamentale per l'economia italiana, la coesione sociale e il presidio del territorio che vanno affrontati e risolti, questo sì, in sede europea. Nel suo piccolo, il disegno di legge che andiamo ad approvare introduce disposizioni a sostegno dell'agricoltura giovanile che vanno oltre quelle dell'autoimprenditorialità; norme che, al contrario di alcune previsioni illogiche europee, possono aiutare a recuperare terre abbandonate e incolte e a valorizzare i beni non utilizzati. Benvenute quindi - lo diciamo con convinzione - le misure che intendono sostenere la competitività delle imprese agricole giovanili e femminili, che andranno inquadrate e finanziate nella nuova politica agricola comune (PAC), che deve implementare ulteriormente il sostegno al ricambio generazionale. I dati ci dicono che le imprese condotte da giovani agricoltori, che sono meno di un decimo del totale, hanno una maggiore redditività e questo va tenuto in considerazione, perché significa che ci sono un impegno, uno studio e un'applicazione anche tecnologica ulteriori rispetto alle attività agricole tradizionali. Ricerca, innovazione e multifunzionalità premiano il lavoro dei giovani agricoltori e sono poi ricompensate dalla loro maggior propensione a investire e innovare anche in attività collaterali all'agricoltura. Insomma, il disegno di legge è incentrato su norme innovative e accompagnato da incentivi fiscali e risorse finanziarie. La stessa strada va seguita a livello europeo, e lo diciamo con convinzione, perché devono essere integrati gli incentivi qui presenti. siamo difensori dell'italianità - tutti dovremmo esserlo e credo che su questo non dovrebbero esserci dubbi - ci teniamo poi anche ad evidenziare che all'interno della nuova PAC devono essere valorizzati i prodotti italiani, che sono unici e non replicabili su altri territori, e che tra l'altro vengono penalizzati anche dal cosiddetto *italian sounding*. Per queste ragioni, con convinzione, sapendo che non si risolvono i problemi certamente solo con questo provvedimento, che

Signor Presidente, signor Sottosegretario, gentili colleghe e colleghi, sappiamo che nel nostro Paese su 740.000 imprese agricole solo più di 100.000 sono gestite È evidente che urge un'attenzione nuova e più corposa per incentivare e agevolare i giovani a intraprendere quello che oggi come non mai appare appare come un lavoro ad altissimo rischio: troppe le perdite che, in congiuntura, possono azzerare il reddito degli agricoltori e per questo, considerando la basilare importanza del settore, è di fondamentale importanza mettere in campo il massimo sforzo per ridurre al minimo perdite che sarebbero insostenibili per qualunque impresa. Fatte queste premesse, arriviamo al disegno di legge sul giovane imprenditore agricolo che stiamo trattando, che si intende volto alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e addirittura al rilancio dell'intero sistema produttivo agricolo, mediante interventi che favorirebbero l'insediamento dei giovani nel settore. Si parla di risorse destinate all'acquisto di terreni e beni strumentali, che giustamente servirebbero, sì, ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni, anche guardando a tecniche di precisione. Benissimo: tutto farebbe pensare dunque che il Governo abbia pensato a grandi investimenti e, quindi, allo stanziamento di cospicue risorse; invece, troviamo solo 15 milioni di euro per tutta Italia

C'è chi dice che è sempre qualcosa e che 15 milioni sono comunque uno stanziamento cospicuo: mi viene allora da collegarmi all'intervento che ha fatto poco fa la collega Floridia riguardo al provvedimento sulla sicurezza del personale scolastico, in cui giustamente, a detta di questa maggioranza, 7 euro a scuola sono qualcosa che può risolvere la problematica. per l'agricoltura dev'essere coperto anche l'altro aiutino inserito nel disegno per i giovani imprenditori agricoli che riguarda chi acquista e permuta terreni agricoli e loro pertinenze: per loro l'imposta di registro, quella ipotecaria e catastale, potrà essere versata nella misura del 60 per cento di quelle previste a legislazione vigente.

un elenco di bellissime proposte, con tante competenze affidate a questo osservatorio, ma sono veri e propri sogni in libertà; rappresentanti del MASAF, il Ministero dell'agricoltura, rappresentanti del Ministero del lavoro, dell'Ismea, dell'Iccrea e associazioni varie, tutti appassionatamente al lavoro per raccolta dati, consulenze, pianificazioni, promozione di politiche attive, politiche di sviluppo rurale, stimoli vari, sostegni e supporti alle più svariate situazioni, dalla formazione, alle fiere, alla creazione di siti Internet; poi giustamente è previsto anche il monitoraggio sull'attuazione di tutte queste misure e la verifica dell'efficacia, per poi proporne modifiche ed integrazioni. C'è tutto, che dire? Un vero e proprio sogno. Ma ci si sveglia subito - e in modo brusco - quando al comma 2 del medesimo articolo è scritto che non ci sarà alcuna copertura, neppure un rimborso spese. Si legge la ormai nota dicitura «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Un applauso davvero per queste soluzioni a costo zero. Penso che solo dormendo si riesca a pensare a ciò. Ci rendiamo conto, quindi, che è una grandiosa presa in giro? Colleghi, davvero credete che questo disegno di legge possa portare un aiuto, che si possa ritenere tale, per i giovani imprenditori agricoli? Vogliamo poi considerare anche le giovani imprenditrici, le donne? Non pervenute. Manca totalmente, nelle politiche di questo Governo, il sostegno alle donne. Nella fase emendativa abbiamo provato a pensarci noi, come MoVimento 5 Stelle, chiedendo che fossero attuate misure per la conciliazione dei molteplici, paralleli e gravosi impegni in ambito familiare assolti dalle donne, agevolandole nel percorso genitoriale. Si parla tanto anche di questo, ma poi nei fatti gli aiuti non ci sono. Sempre per questo fondamentale aspetto abbiamo proposto un incremento del fondo per l'imprenditoria femminile in agricoltura e abbiamo preteso una considerazione speciale per la tutela della genitorialità, quando si parla di servizi di sostituzione nell'azienda agricola. Sapete cosa è successo? Nulla, perché l'argomento non interessa alla maggioranza, troppo presa a dover chiudere il testo, sempre di corsa; un testo che però rimarrà in un cassetto, senza produrre effetti di rilievo. È un altro inutile tassello, che andrà ad aggiungersi al castello di carta di promesse vuote, purtroppo, di questo Governo. Come dicevo, noi abbiamo provato a tracciare, con i nostri emendamenti, l'idea di imprenditoria giovanile agricola e lo abbiamo fatto recependo le richieste che il comparto avanza da anni. Le viviamo anche giornalmente, nei vari presidi, presidi, dove vado ad ascoltarli direttamente. Forse, invece, questo Governo è troppo lontano dalla strada, dove si riuniscono gli agricoltori per far valere la propria voce. Parlo prima di tutto della stabilizzazione degli sgravi contributivi e del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali. E ancora, in un momento in cui le imprese sono sferzate da rincari *record*, che portano alle stelle i costi di produzione, noi abbiamo richiesto una moratoria al credito, con una sospensione per dodici mesi del pagamento di rate e canoni, per dare una boccata di ossigeno a tutte le aziende che davvero rischiano di indebitarsi a dismisura, in attesa attesa di poter avere un raccolto utile. Abbiamo messo in campo proposte per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico delle imprese giovanili nell'agricoltura, ma anche per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari e per le aree interne e marginali. Non abbiamo poi dimenticato un altro aspetto fondamentale, quello del recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico, attraverso l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali: una vera ricchezza che abbiamo nella nostra varietà italiana. È una questione, quest'ultima, su cui l'Esecutivo continua ad indugiare, perché tirato per la giacca dalle prerogative di una Lega che guarda sempre troppo al Nord, senza tener conto del fatto che c'è un Sud che crea utili e deve essere supportato in questo processo. *(Applausi)*. Riequilibrare le forze e distribuire equamente i soldi: queste devono essere le parole d'ordine. Ma dietro la barriera delle cosiddette scelte politiche, la Meloni continua a distribuire le risorse in maniera iniqua, introducendo sistemi regressivi in cui i più ricchi pagano meno. Servirebbe invece combattere con reale impegno l'evasione fiscale per coprire le misure vere che l'Italia sta aspettando. Quando ci viene detto che non ci sono le risorse per investire in ospedali, in personale medico, negli insegnanti, in scuole sicure e anche per prorogare l'Irpef agricola al 100 per cento, il Governo sta mentendo; i soldi ci sono, basterebbe che tutti versassero le imposte e si andasse a pescare tra gli extraprofitti. Lo diciamo da sempre, come MoVimento 5 Stelle: gli extraprofitti vanno attaccati. legge è solo un flebile atto di indirizzo generale, una sorta di politica di indirizzo, ma il vento sta cambiando e le prime avvisaglie della rivolta degli onesti ce le ha date la vittoria in Sardegna della nostra Alessandra Todde. Quindi, parlare in un disegno di legge di politica di indirizzo non porta a terra nulla, nulla di concreto e tutto resta campato in aria. Sogni in libertà, come ho detto all'inizio; concedersi la libertà di sognare a occhi aperti è una cosa meravigliosa e può rendere sereno chi però non vive sulla sua pelle i reali problemi. Per loro serve concretezza. Il voto del MoVimento 5 Stelle sarà di astensione solo in riferimento alle tante belle parole spese in questo provvedimento. Più che un disegno di legge, ha l'aspetto di un ordine del giorno con degli impegni al Governo. Ed è proprio per quegli impegni che non diamo il voto contrario, ma è a quegli impegni che è doveroso riportare riportare questa maggioranza. difendere l'agricoltura italiana, che è la migliore agricoltura al mondo, difendere il *made in Italy* e difendere i prodotti della nostra terra è la nostra missione e deve essere la missione di tutti i partiti e di tutta la politica italiana. Un Paese senza agricoltura è un Paese che non ha futuro *(Applausi)*, come giustamente ci ricordano gli agricoltori che in questi giorni scendono in piazza contro le folli politiche dell'Europa. dell'Europa. Ancora una volta, tocca allora a noi della Lega raccogliere le istanze degli agricoltori italiani e promuovere questo disegno di legge che ha l'obiettivo di aiutare concretamente i giovani agricoltori, fornendo loro gli strumenti necessari per iniziare un'attività nel settore agricolo. Questo provvedimento è un messaggio di speranza rivolto ai nostri giovani, perché pone l'attenzione sul grande tema del ricambio generazionale, che rappresenta una sfida fondamentale per il futuro dell'agricoltura italiana; un ricambio generazionale che nel nostro Paese è particolarmente difficile, ma assolutamente necessario, considerato che soltanto il 9 per cento delle aziende agricole è guidato da giovani. Se l'Italia vuole continuare ad avere la migliore agricoltura al mondo, deve necessariamente investire sui giovani. Se l'Italia vuole continuare ad essere la numero uno al mondo nel settore dell'agroalimentare, deve favorire il ricambio generazionale e aiutare i nostri giovani a scendere in campo. *(Applausi)*. Dobbiamo dire a voce alta fare il contadino nel 2024 significa innovazione, specializzazione, formazione di alta qualità, non soltanto agricola, ma anche commerciale e finanziaria. Fare l'agricoltore al giorno d'oggi significa conoscere e utilizzare tecnologie di ultima generazione, ricerca scientifica e nanotecnologie. Il tutto, ovviamente, è coniugato con i saperi e le tradizioni che abbiamo ereditato dai nostri padri e che fanno del *made in Italy* un patrimonio unico al mondo. Solo se sapremo unire tradizione e innovazione, passato e futuro, saremo in grado di difendere veramente il *made in Italy* e rendere più competitive le nostre aziende. Tutti noi abbiamo il dovere di credere nella gioventù agricola e lo dobbiamo fare con leggi come questa, che introducono misure necessarie e di buon senso, come il taglio della burocrazia, la facilità di accesso al credito e una serie di esenzioni e agevolazioni fiscali per l'acquisto dei terreni e dei primi insediamenti. Se vogliamo dare un futuro all'agricoltura italiana, la prima, vera questione da affrontare è la sostenibilità economica delle nostre aziende agricole. Dobbiamo ribaltare il falso paradigma portato avanti dai burocrati europei e dalla sinistra italiana, perché la redditività delle imprese viene prima di tutto. La sostenibilità ambientale non si realizzerà mai se prima non vengono tutelate e garantite la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale delle nostre imprese, dei nostri lavoratori e delle nostre famiglie. Da settimane stiamo assistendo alle giuste proteste degli agricoltori che si stanno ribellando contro le politiche scellerate dell'Europa che rischiano di distruggere il sistema agroalimentare italiano. In questi anni a Roma, e soprattutto a Bruxelles, la Lega è sempre stata in prima fila, spesso da sola, nella battaglia per fermare *(Applausi)* regolamenti e direttive europee che avrebbero fatto chiudere migliaia di aziende agricole italiane. Grazie alla Lega, in questi mesi di Governo di centrodestra, abbiamo portato a casa risultati importanti per l'agricoltura italiana. Pensiamo a questa legge sulla gioventù agricola, agricola, alla legge sull'agricoltore custode dell'ambiente, all'esenzione Irpef per i redditi agricoli dominicali che è stata reintrodotta grazie alla battaglia della Lega. Noi saremo sempre a fianco degli agricoltori. Noi saremo sempre dalla parte di chi lavora e di chi produce, dalla parte di chi lotta ogni giorno per difendere il *made in Italy* e l'agricoltura italiana. Per questi motivi, signor Presidente, annuncio con orgoglio il volto favorevole del Gruppo Lega Salvini-*Premier*. esame è valutato cardine dall'Agenda europea, è un punto di forza di quello che è il piano strategico della PAC. È un provvedimento che si pone lo scopo di generare un ricambio generazionale in un settore estremamente difficile e in difficoltà come l'agricoltura. È un provvedimento sul primo insediamento, quello che solitamente viene definito, definito, ed è strategico anche per i motivi rilevati dagli illustri colleghi e colleghe negli interventi precedenti. Noi abbiamo un sistema delle imprese agricole che vede solo un 10 per cento di imprese in mano a giovani agricoltori. È un dato che è diminuito di molti punti percentuali negli ultimi dieci anni e, così proseguendo le politiche, è destinato ulteriormente ad impoverirsi. Impoverire il ricambio generazionale vuol dire vanificare tutto quello che noi diciamo del *made in Italy*, delle nostre produzioni; rendere più difficile la custodia dei nostri territori, molto spesso aree interne. cento del nostro Paese sono aree interne che, senza un'attività agricola di presidio, di tutela e di salvaguardia, rischiano di produrre effetti negativi, come dico sempre, a valle. Quando infatti si verifica un grave evento calamitoso, parte dalla montagna e dalle colline e si riversa nelle aree più antropizzate che si trovano a valle. Noi abbiamo dato il sostegno ad un provvedimento che è quello dell'agricoltore custode, perché noi riteniamo che non esiste agricoltore senza ambiente, non esiste ambiente senza agricoltore

È l'agricoltore il primo che subisce gli effetti del cambiamento climatico, perché le sue attività sono in campo aperto, non sono sotto il tetto di un capannone. E, ogni qual volta interviene un fenomeno, è lui che ne subisce gli effetti in via principale. Le imprese agricole giovanili sono 60.000 al Sud, 16.000 al Centro e 30.000 al Nord. La maggioranza dei terreni è al Sud. Noi, pur condividendo il principio che l'Europa ci dice in merito al ricambio generazionale come punto cardine del piano strategico della PAC, non possiamo dare un voto favorevole a questo provvedimento, per il metodo che è stato utilizzato. un metodo sbagliato, perché questo provvedimento non ha un colore politico, ma risponde a un'esigenza economico-sociale di salvaguardia dell'agricoltura. Su questo si rendeva necessario che quel percorso iniziato in Commissione parlamentare alla Camera, che aveva visto molta condivisione, non fosse stralciato all'ultimo momento. Il nostro no a questo provvedimento nasce prevalentemente dal metodo e dai suoi contenuti economici. *(Applausi)*. Qualcuno ha detto che non ci si può astenere su un provvedimento o votare contro un provvedimento che favorisce il ricambio generazionale. Ma noi non ce la sentiamo di prendere in giro gli agricoltori, dicendo loro che con 15 milioni di euro su tutto il territorio nazionale risolviamo i problemi dell'agricoltura giovanile. Non ci possiamo permettere, in un momento in cui le aziende agricole stanno soffrendo, di dire loro che noi oggi votiamo un titolo, ma non i suoi contenuti. Abbiamo bisogno di dare risposte concrete e non possiamo essere visti come quelli che parlano e parlano, ma che poi non producono fatti sufficienti per

perché, se gli agricoltori spopoleranno quelle aree, ci troveremo in difficoltà ancor più gravi di quelle che siamo chiamati a fronteggiare giornalmente. Mi spiace dirlo,

Quell'emendamento era stato proposto in legge di bilancio e non se ne è voluto discutere, per un approccio che talvolta appare estremamente arrogante - scusate il termine - nell'affrontare le questioni, in assenza di confronto. Cosa che devo dire, per onestà intellettuale, è diversa rispetto a quello che avviene nella nostra Commissione, in cui, partendo da posizioni diverse, si dialoga, si discute e si fa ogni sforzo per cercare di andare incontro ad esigenze di buon senso.

Del pari in legge di bilancio non si è rinnovata un'altra misura, l'esonero contributivo e la decontribuzione INPS per i giovani agricoltori, che vale 2.000-3.000 euro ad azienda. poca cosa a parlarne, ma, per chi deve svolgere un'attività con una marginalità che ormai oggi è inesistente, è un'altra piccola misura. Non si risolvono i problemi dell'agricoltura con un colpo di genio, purtroppo, ma con tante piccole misure che, sommate l'una all'altra, possono dare ai giovani agricoltori quello spirito che trasmettono loro i propri padri e le proprie madri e che li spinge a continuare un mestiere che oggi si presenta sempre più difficile.

sugli acquisti e tutta una serie di piccole misure che avrebbero aiutato un giovane ad approcciarsi a questa attività, che è estremamente complessa. Potremmo dilungarci molto sui vari temi, ma il vero elemento essenziale ed ultimo è un altro: da un lato si sbandiera l'autonomia differenziata; dall'altro lato si centralizza, con un provvedimento del Ministero, la definizione dei criteri di assegnazione su base nazionale

la capacità di definire i criteri cardine, perno su cui poi dare questi pochi e modesti incentivi, che onestamente sono totalmente irrisori, avvenisse su base regionale. Questa contraddittorietà continua rende l'idea di un Governo confuso nell'assunzione dei provvedimenti: provvedimenti presi all'ultimo minuto, provvedimenti presi di corsa, provvedimenti che mortificano anche l'attività parlamentare, che dovrebbe essere di confronto, di discussione e di sintesi, quantomeno su provvedimenti come questi. Provvedimenti che non hanno una identità etica, perché credo che qui nessuno possa dire che è sbagliato dare un contributo, per il ricambio generazionale e per l'incentivo a giovani donne e giovani uomini che si vogliono approcciare a questo mestiere.

a me corre l'obbligo di chiudere questo dibattito, a volte abbastanza stucchevole, rispetto ai temi dell'agricoltura, non come quello studente

Probabilmente, qualcuno lavora meglio da dormiente di qualcun altro da sveglio. *(Applausi)*. Questo è palese ed evidente anche quando parliamo degli ultimi vent'anni della storia dell'agricoltura nazionale e europea. In vent'anni, l'Europa, con la complicità delle forze politiche che hanno governato questa Nazione, ha destinato un terzo delle risorse comunitarie a diminuire la produzione, non ad aumentarla. *(Applausi)*. Una PAC che nasceva con lo scopo di con lo scopo di garantire gli approvvigionamenti e sostenere il reddito degli agricoltori si è trasformata, negli anni, da forte sostegno anche alla multifunzionalità (che è quella che oggi fa stare in piedi

dimostrazioni di quanto sia fallimentare questa politica si hanno oggi con le manifestazioni in piazza. A tutto questo abbiamo dato concretamente delle risposte, che sono, appunto, tangibili. Una di queste è contenuta in questa manovra, che è una manovra, sì, di sostegno ai giovani. È vero, noi abbiamo un *gap* rispetto ai giovani delle altre Nazioni, ma qui mi corre l'obbligo

il mio omologo della Camera, onorevole Carloni. Ma sappiamo benissimo che questa è la cornice all'interno della quale possiamo costruire una nuova visione dell'agricoltura, che veda il giovane protagonista, proprio per la sua straordinaria capacità di fare innovazione, di un approccio verso l'agricoltura che non punti alla decrescita, posto che qualcuno la definisce addirittura decrescita felice. Io non ho mai visto nessuno decrescere felicemente. Ho visto solo gente decrescere in maniera infelice, ma questa è un'altra partita. Sono altri i partiti che perorano queste visioni. Noi abbiamo una visione diversa, che è quella per cui, attraverso l'innovazione, attraverso la ricerca, attraverso lo studio e l'applicazione, non con le enunciazioni di semplici *slogan*, potremo affrontare temi delicati, come quello del cambiamento climatico, con strumenti aggiornati e moderni, che ci consentono di avere un'agricoltura che riesca a mantenere e perpetrare la straordinaria tradizione di cui godiamo.

regionale all'interno di questo *record* nazionale di DOP e di IGP, a dimostrazione di un valore aggiunto riconosciuto non solo in Italia ma anche all'estero, su cui

un bagaglio culturale anche sotto il profilo dell'agroalimentare che ci permette di affrontare il mondo con una certa fiducia. In questi giorni ho incontrato dei giovani: ne cito tre, perché mi

che la politica agricola comune (PAC) così com'è non funziona e che porta delle proposte che non si limitano alle proteste, ma che costituiscono una piattaforma su cui far lavorare e far convergere anche altri Paesi che fino a oggi sono stati succubi di una politica straordinariamente bieca e cieca,

che se oggi non c'è il passaggio generazionale tra i genitori e i figli, è solamente perché i genitori disincentivano i figli a fare quel lavoro se non ha remunerazione e redditività. Questa è la partita su cui dobbiamo intervenire, non sulle filosofie come il *green* che hanno

che ci sono attività, come quella agricola, che non constano solo di una mera produzione di prodotti, anche se questo dovrebbe bastare. Infatti, chi oggi si appella alla riduzione di tutto ciò che potrebbe essere convenzionale, dimentica di ricordare che, se non vogliamo abbandonarci al destino di mangiare

L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1020 recante: «Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali», Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali". Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577,

571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni appaiono quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica». Grazie